a condizione che fossero approvate alcune modifiche. Chiedo ai presentatori se intendono accogliere le proposte di modifica avanzate dal ministro della salute, professor Fazio.

una rinnovata volontà del Governo di andare oltre, per alcuni versi, rispetto alla richiesta formulata nella mozione, anzi, hanno sottoposto la necessità di fare un passo in avanti. Il Governo in quella direzione si è già mosso e intende muoversi con maggiore e più incisiva determinazione. Questo è apprezzabile e, pertanto, la condivisione è solidamente appoggiata su questa considerazione.

onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, è stato detto tutto ieri, in una discussione effettivamente molto ricca. Io sono grato alla senatrice Soliani, che ha consentito che io apponessi la mia firma alla sua mozione e ai colleghi che hanno

in qualche modo, un problema delle famiglie, che oggi rispondono a molte delle incertezze che il sistema rivela intorno a questa patologia. La demografia ci sta dicendo che tra qualche tempo queste famiglie non saranno più così come noi le immaginiamo. Saranno moltissimi gli anziani soli soli e, a quel punto, il sistema dovrà dare una risposta, che soltanto se viene preparata oggi potrà essere adeguata. Per questo motivo, in quelle mozioni si chiede una tensione educativa, soprattutto nei confronti dei medici di famiglia, che per primi oggi, e forse unici domani, potranno cogliere gli scricchiolii di quella memoria che va via e che ci rende interessanti, perché ci fa unici. Se i medici cogliessero in questo modello l'opportunità di una passione nuova per il loro antico mestiere, quello della relazione con la persona, questo tempo di discussione dentro un'Aula parlamentare avrebbe avuto anche un suo significato. Così come servirebbe dare da subito una risposta integrata tra il sanitario e il sociale per creare un punto di accesso che non renda il familiare un vagabondo tra le diverse strutture e per capire quel che deve fare.

Sappiamo che le emozioni qualche volta valgono un battito d'ali: speriamo che queste aiutino. Come diceva molto bene il senatore Bosone ieri, se l'Alzheimer non è una sconfinata giovinezza, almeno cerchiamo di fare in modo che non sia uno sconfinato dolore.

che i periodi di crisi, a cui ormai siamo abituati - come hanno ricordato anche i relatori prima di me - non vadano ad inficiare o a compromettere gli stanziamenti necessari per combattere adeguatamente questa malattia. Sono convinto che, facendo bene il conto della spesa e mettendo sul piatto della bilancia il rapporto costi-benefici, il minimo investimento che dovrà essere stanziato a protezione di questa malattia farà risparmiare sicuramente

come ricordava anche la senatrice Garavaglia - perché molti di noi hanno visto da vicino, in famiglia o tra gli amici, cosa significa essere ammalati di

determinando nel malato un lento e graduale deterioramento delle capacità cognitive: la memoria, l'attenzione, il linguaggio, il pensiero

e un'attenzione più generale della comunità. Pertanto, questa malattia diventa una graduale discesa all'inferno, non solo per il malato, ma anche per i familiari, che soffrono per il carico di fatica

per chi oggi invece ha bisogno di essere assistito e di vedere riconosciuta la propria malattia. Per questo motivo, ringraziando la senatrice Soliani che si è fatta promotrice

Colgo l'occasione per ringraziare la Presidenza del Senato, che mesi or sono ha dimostrato una grande sensibilità nei confronti di questa patologia, permettendo, per la prima volta, in sala Zuccari, la proiezione di un film, dal titolo «Una sconfinata giovinezza»,

per la salute e la promozione del diritto alla prevenzione, vide la commossa partecipazione del ministro Fazio, che voglio ringraziare per la sua esposizione, nella replica di ieri, dei 10 punti programmatici,

La proposta della Commissione, tra gli altri punti, prevede anche l'abrogazione del regolamento 41/2009/CE, relativo

intende porre di fronte al Governo le pesanti ripercussioni che l'abrogazione di tale normativa produrrebbe a carico dei tanti celiaci, che ad oggi nel nostro Paese possono invece contare su una legislazione che tutela la loro salute e li rende consapevoli della pericolosità di contaminazione. L'intolleranza al glutine, infatti, causa gravi lesioni alla mucosa dell'intestino tenue, che regrediscono eliminando il glutine dalla dieta. La reversibilità della patologia è strettamente legata alla non assunzione da parte del soggetto celiaco di alimenti contenenti glutine o comunque da esso contaminati. Il soggetto celiaco è affetto da una malattia cronica, non guarisce purtroppo, ma rimane tale per tutta la sua vita. L'unica - ripeto l'unica - cura consiste nell'adozione di una dieta rigorosamente priva di glutine. Siamo in presenza di una patologia largamente diffusa e non è certamente un caso che l'articolo 1 della legge n. 123 del 2005 la riconosca come una «malattia sociale». Tale legge - lo ricordo perché ero presente in quella legislatura - fu approvata all'unanimità dall'Aula e ha fatto sì che l'Italia adottasse un provvedimento di alta civiltà, che è stato anche di esempio per altri Paesi. Stime accreditate dimostrano come in Italia i potenziali celiaci siano circa 600.000, quelli diagnosticati circa 60.000 e, ogni anno, sono circa 2.800 i nuovi casi che vengono diagnosticati. Ma non è una situazione confinata al nostro Paese. La celiachia è considerata una patologia diffusa in maniera omogenea a livello mondiale, anche se presenta una più elevata incidenza proprio in Europa, nel Vecchio continente. Questi numeri fanno della celiachia la più frequente intolleranza alimentare a livello globale. Allo stato attuale i prodotti senza glutine vengono considerati prodotti dietetici e garantiscono totale sicurezza per il consumatore celiaco. Nel nostro Paese, inoltre, tali prodotti sono elencati nel cosiddetto registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine (come da decreto legislativo n. 111 del 1992) e vengono erogati gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale in forza della legge n. 123 del 2005. È dunque un segnale importante e positivo la rapidissima calendarizzazione di questa mozione - di questo ringrazio il Presidente e la Conferenza dei Capigruppo

un esito peraltro auspicato dalle tante associazioni dei pazienti presenti nel nostro Paese, che attendono con speranza il voto di oggi, ma anche dai produttori di prodotti per celiaci. La mozione al nostro esame prende atto e recepisce l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione sanità e dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea. Entrambe le Commissioni hanno espresso netta contrarietà con riferimento alle norme applicabili ai prodotti per celiaci, sia con riguardo alla violazione del principio di proporzionalità e di sussidiarietà di matrice comunitaria. In particolare, pur condividendo l'obiettivo di armonizzazione perseguito dalla Commissione europea, volto ad un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, si è convenuto che la proposta di abrogazione non tiene conto in maniera sufficiente delle «esigenze connesse con la tutela della salute umana», così come imposto dall'articolo 9 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Come è stato correttamente osservato dalle Commissioni 12a e 14a, la distinzione tra persone sane e persone che hanno problemi di salute impone per forza di cose la necessità di una regolamentazione differente. Per le prime può valere la disciplina generica di tutela del consumatore, senza che ciò comporti pregiudizi di sorta; per le seconde occorre, invece, una disciplina specifica che tuteli la loro condizione fisica. Situazioni diverse devono essere disciplinate in modo differente in un'ottica di garanzie di parità di trattamento. Nel caso al nostro esame esiste già una disciplina specifica, quella di cui al citato regolamento della Comunità europea n. 41 del 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari

Commissione europea appare debole anche da un punto di vista squisitamente giuridico e non sarebbe giustificata, né in un'ottica di proporzionalità, né in un'ottica di sussidiarietà. Come osservato dalle Commissioni 12a e 14a, non si ravvisa, infatti, la necessità di procedere all'abrogazione di un regolamento comunitario che reca, al contrario, una disciplina necessaria, che soddisfa pienamente le esigenze dei pazienti. L'eliminazione dal mondo giuridico di questa normativa implicherebbe, infatti, un evidente arretramento della tutela delle persone affette da celiachia, anche rispetto agli elevati *standard* di salvaguardia previsti dall'ordinamento italiano, che tutela i bambini e gli adulti come categoria di consumatori vulnerabili. Vi è poi un altro aspetto da segnalare. L'abrogazione del concetto di «prodotto dietetico», e la conseguente equiparazione dei prodotti senza glutine

di ottenere il rimborso di questi prodotti da parte del Servizio sanitario nazionale e la conseguente necessità di rivisitare - stante la prevalenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno tutta la normativa di maggior tutela per le persone affette da celiachia o altra malattia socialmente rilevante. Allora, una domanda nasce spontanea: è davvero necessario tutto questo? Per ragioni giuridiche, oltre che di buon senso, la risposta è certamente negativa. L'esigenza di semplificazione perseguita dall'Unione Europea deve cedere il passo di fronte ai diritti fondamentali della persona che sono, per loro natura, incomprimibili, soprattutto laddove come nel caso che stiamo analizzando - ciò comporta l'indebolimento delle tutele fino ad oggi garantite ai soggetti celiaci, e in ordine alle quali si è già consolidato un legittimo affidamento. La presenza di interessi sensibili di rango primario determina l'impraticabilità dei modelli di semplificazione. Si tratta di un principio consolidato ed è la bussola che guida l'azione dei pubblici poteri. Come è possibile parlare di diritto comunitario che lede il diritto della persona? Peraltro, la tanto auspicata semplificazione rischierebbe, di fatto, di sortire - le chiedo un minuto in più, Presidente Presidente - proprio l'effetto opposto, perché innescherebbe nel nostro ordinamento un procedimento di revisione della normativa relativa alla commercializzazione dei prodotti senza glutine e al regime di rimborsabilità degli alimenti. Concludendo, mi permetto di affermare che forse sono troppo i disagi che la proposta della Commissione europea introduce, sia per il nostro Paese che per gli altri Paesi europei. L'impegno contenuto nella mozione è quello di promuovere, in sede comunitaria e nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le iniziative necessarie al fine di tutelare una categoria di cittadini sensibili, come i celiaci, dai rischi alla salute connessi all'abrogazione del regolamento

che non parte dalla tutela della salute sia un'Europa che facciamo fatica ad amare.

semplificazione, innovazione e armonizzazione fanno rima con garanzia e tutela, e il problema è proprio questo: la proposta

determina non marginali profili di pregiudizio per la tutela della salute pubblica. sostanzialmente il regolamento introduce disposizioni innovative in materia di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e di alimenti destinati a fini medici speciali. - ed è questo il punto di discussione, tra l'altro - l'abolizione del regolamento n. 41 del 2009, che sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2012. Questo viene proposto dalla Commissione europea al fine di creare una procedura semplificata che - ritiene la stessa Commissione - interpreti l'esigenza di armonizzare le legislazioni dei Paesi membri e consenta la migliore e più adeguata circolazione delle merci garantendo maggiormente le esigenze del cittadino consumatore. Non è assolutamente così, perché questo processo di presunta semplificazione arreca danno ad un

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative si conclude stabilendo che in particolare in materia di sanità e di protezione dei consumatori la Commissione europea nelle sue proposte si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Orbene, l'approvazione, così come vorrebbe la Commissione di un regolamento che spazza via il regolamento n. 41 di fatto determina un terremoto nell'ambito della legislazione domestica, con particolare riferimento a quanto nel nostro Paese da oltre trent'anni e in modo assolutamente puntuale è stato fatto sul versante della tutela delle esigenze e dei diritti e della protezione non soltanto sanitaria del paziente celiaco: celiaco: oltre trent'anni di legislazione domestica orientata in tale direzione, che trova riscontro in provvedimenti che partono dal 1953 e accompagnano un percorso che evolve con normative anche di rango europeo, in particolare quella del 1977, che approdano nella nota e più volte citata legge n. 123 del 2005 che porta il titolo «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia», là dove si dice che gli interventi riferiti a questa legge, unitamente agli interventi generali di servizio sanitario, sono finalizzati a favorire a favorire l'inserimento nella vita sociale dei pazienti affetti da celiachia con oneri a carico del Servizio sanitario.

Il pronunziamento complessivo e unanime è stato inequivocabile e incontrovertibile, senza se e senza ma: un no secco e deciso ad un un momento di distrazione, chiamiamolo così, ma se vogliamo essere un po' più precisi forse dovremmo dire ad un maldestro tentativo di far prevalere, come talvolta accade, la cultura del mercato che viene propugnata dietro la bandiera del cosiddetto mercatismo dai profeti della primazia

sentinelle attente e accorte anche in quest'Aula, dove noi tutti, interpreti del nostro ruolo, ci schieriamo come paladini delle esigenze della comunità e in particolare di una fascia di soggetti deboli, che oggi trovano una normativa adeguata e che addirittura potrebbe ulteriormente progredire in termini di livelli di protezione ma che già oggi è sufficiente, che non è possibile non è possibile fessurare in nessun punto e non è possibile vulnerare per tentare di aprirvi una scorciatoia per far entrare chissà quale principio non certamente condivisibile rispetto alle esigenze che vogliamo sostenere. In Italia i prodotti per celiaci sono controllati; chi li fabbrica è vigilato dal Ministero della salute,

e conseguentemente conservare, attraverso la preservazione del regolamento n. 41 del 2009, quel famoso registro registro in cui sono indicati i pazienti affetti da celiachia, che hanno diritto ad avere i prodotti alimentari adatti alla loro dieta con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Se in Europa dovesse passare questa direttiva, indubbiamente noi faremmo un passo indietro. So che non lo vuol fare l'Italia; so che il Parlamento esprimerà anche oggi una rinnovata ed inequivocabile posizione in tal senso. So che il Ministro della salute, per l'autorevolezza personale, per l'impegno profuso ed anche per il ruolo di rappresentanza che in sede comunitaria svolge a nome del Governo, non soltanto ribadirà un secco no ma saprà creare momenti di aggregazione attorno a questo principio con altri Paesi dell'Unione, per ergere una diga che eviti di aprire un declino perverso e di grave pregiudizio per il lavoro che in tanti anni, in più legislature, Governi di tutti i colori hanno realizzato per dare una risposta ad una platea di soggetti fragili, che deve essere ancora tutelata e che non può essere esposta a rischi di alcun genere. Ringrazio il Ministro per il suo impegno e per quanto vorrà fare a sostegno delle tesi che anche oggi in quest'Aula sono state esposte. Signor Presidente, Ministro, colleghi senatori, la Commissione europea, il 20 giugno di quest'anno, ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati ai fini medici fini medici speciali. Con questa proposta, essa intende rivedere le disposizioni in materia di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare contenute nella direttiva 2009/39/CE, designata come «Direttiva quadro sui prodotti dietetici». Lo scopo di questa proposta di regolamento dal punto di vista della Commissione è quello di armonizzare, semplificare ed aggiornare le norme applicabili alla composizione e all'etichettatura di categorie specifiche di alimenti, con l'obiettivo di fornire ai consumatori prodotti adeguati sotto il profilo nutrizionale,

del regolamento (CE) n. 1924/2006, destinato alla commercializzazione ed etichettatura dei prodotti alimentari ad uso corrente con la conseguente equiparazione; tale intervento riguarderebbe un'ampia categoria di prodotti destinati a chi è affetto da celiachia e che ha, quindi, la necessità di eliminare totalmente e per tutta la vita il glutine dalla propria dieta; i celiaci sono una categoria sensibile di consumatori poiché la celiachia è un'intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale. Attualmente in Italia risulta affetta da celiachia una persona su 100, e l'intervento della Commissione europea, anche se volto a semplificare la vita la vita al consumatore generico, rischia invece di complicarla ad alcune categorie vulnerabili di cittadini, come appunto i celiaci, riducendo le garanzie di sicurezza dei prodotti dietetici senza glutine, che attualmente sono sottoposti al regime di notifica su tutto il territorio europeo:

se verrà adottata dalla Commissione e dall'Europa, è di cancellare la definizione di «prodotto dietetico» e di ridurre la dicitura «senza glutine» ad un'etichetta generica. Di fatto si andrà ad abrogare il registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine (previsto dal decreto legislativo n. 111 del 1992), che rappresenta un sostegno fondamentale ai celiaci, in quanto raccoglie i prodotti erogabili a carico del Sistema sanitario nazionale. Pertanto, la proposta della Commissione abolisce il concetto di alimenti dietetici e istituisce un nuovo quadro, contenente disposizioni generali soltanto per un numero limitato di categorie ben definite di alimenti, giudicati essenziali solo per alcuni gruppi vulnerabili della popolazione: in questo caso, alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti da utilizzare sotto la sorveglianza di un medico. la distinzione tra persone sane e persone che hanno problemi di salute impone una differenza di disciplina. Per le prime può valere la disciplina generica di tutela del consumatore, per le seconde occorre una disciplina specifica che, per le persone affette da celiachia come nel caso di specie, appare già correttamente individuata, appunto, nel regolamento 41/2009/CE che si intende abrogare. Ne consegue che abrogando detto regolamento si corre il rischio di un arretramento il rischio di un arretramento sostanziale nella tutela delle persone affette da celiachia. Le esigenze di tutela della salute dovrebbero comportare non solo di mantenere la vigenza del regolamento (CE) n. 41/2009, ma anche eventualmente di elevarne il rango nell'ambito delle fonti del diritto dell'Unione europea;

Commissione europea, prevede l'abrogazione della direttiva n. 8 del 1996 che riguarda le persone affette da obesità e da sovrappeso. La Commissione sanità ritiene anche necessario un supplemento di riflessione sull'esclusione sull'esclusione delle persone in sovrappeso dalla categoria dei gruppi vulnerabili della popolazione, cui la proposta di direttiva reca una disciplina specifica. L'Organizzazione mondiale della sanità reputa infatti che il sovrappeso e l'obesità siano tra i fattori di maggior rischio per un numero rilevante di malattie croniche,

Signor Presidente, il Governo accoglie integralmente e senza riformulazioni le tre mozioni presentate. Vorrei garantire agli onorevoli senatori il massimo impegno

delicatezza della materia che stiamo trattando oggi. La stessa mia firma alla mozione della senatrice Baio testimonia la comune sensibilità dei colleghi senatori dell'Italia dei Valori

signor Ministro, la legge n. 123 del 2005 prevede che annualmente il Ministro della sanità riferisca al Parlamento sulla situazione in termini di monitoraggio e di stato dell'arte della malattia celiaca. Ora, se lei rivede le sue relazioni, in modo particolare quelle del 2008 e del 2009, esse hanno in comune due aspetti che devono richiamare un po' la nostra attenzione. In primo luogo, queste relazioni dicono che dal momento della comparsa dei sintomi al momento della diagnosi della malattia celiaca intercorre un periodo medio di sei anni.

nei confronti delle nostre popolazioni, perché molto spesso l'astenia, che è il pre-sintomo della malattia celiaca, viene identificata genericamente, con diagnosi sbagliate. Il secondo aspetto di queste relazioni annuali che lei, Ministro, ha fornito puntualmente al Parlamento che per ogni diagnosi di malattia celiaca che viene fatta ve ne sono dieci che mancano, per cui, in realtà, i pazienti, quantificati in circa 60.000, come è stato ricordato, sono

sull'esatta quantificazione dello sforzo che la politica sanitaria nazionale e le politiche sanitarie regionali devono fare in questo campo. Ma non è solo una questione di una platea decisamente più ampia e complessa: lei mi insegna anche che le complicanze dovute ad un'errata diagnosi o ad una diagnosi non fatta sono pesanti; lo stesso suo rapporto annuale fa riferimento a possibili

a qualche riflessione sulla copertura economica di cui ha usufruito la legge n. 123. Lei sa, signor Ministro, che la copertura economica di questa legge, che riguarda una malattia sociale che tutti hanno ricordato come una delle più importanti

Dico questo anche perché, signor Ministro, non basta una buona legge, ma occorre anche che da parte del Ministero che lei dirige vi sia anche un attento monitoraggio di questa legge.

vi sono diverse Regioni, soprattutto del Sud, che hanno livelli di adeguamento assolutamente bassi e improponibili. Dico queste cose non per polemica, perché né la seduta né il momento ci ci invitano a fare polemiche di qualsiasi genere, ma semplicemente perché ci rendiamo conto che la nostra coscienza sarà realmente a posto non solo quando approveremo all'unanimità le singole mozioni, ma quando poi ci sarà da parte del Governo e del Parlamento un attento e capillare monitoraggio delle cose che approviamo. Detto questo, sottolineo che i colleghi che hanno in maniera approfondita illustrato la proposta di regolamento europeo COM 353 sono stati di una sobrietà più unica che rara, perché questa proposta di regolamento grida vendetta. grida vendetta. Ho quindi apprezzato la vostra sobrietà di toni, così come ho apprezzato anche la risoluzione che è stata votata dalla 12a Commissione, che invito il Ministro a leggere, o a rileggere, perché è estremamente esaustiva

che per certi aspetti è molto più avanti rispetto ai principi che tuteliamo noi come Parlamento italiano. Noi parliamo, infatti, di livelli essenziali di assistenza;

Signor Ministro, voglio esserle di aiuto nel sottolineare come questa proposta sia assolutamente ribaltabile, perché nelle premesse della relazione ci sono due punti di assoluta inconsistenza.

l'applicazione del vasto concetto dei progetti alimentari, su cui è basata questa direttiva, comporta problemi per gli operatori interessati e per le autorità di sorveglianza». Non parla di pazienti, ma di operatori interessati e di autorità di sorveglianza. Fanno un'ulteriore frittata perché, sebbene sia riconosciuta l'utilità di mantenere in vigore le norme di talune specifiche categorie di prodotti alimentari, correlati a benefici nutrizionali, la necessità dell'esistenza di una siffatta categoria di prodotti alimentari è ancora messa in seria discussione.

Signor Ministro, il Governo ha tutte le armi a disposizione per poter fare in modo che la proposta COM 353 venga eliminata,

possono essere revocati dal Consiglio e dal Parlamento europeo entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea.

non è soltanto in carico al Governo e al Ministro della salute, ma è in carico a tutto il Parlamento nazionale italiano, che deve farsi carico, presso i propri Gruppi in Europa, per fare in modo di applicare immediatamente

mi ostino a voler imparare qualcosa e posso riflettere sul fatto che, quando la semplificazione avviene ad ogni costo e finisce per complicare la vita dei più fragili, diventa una semplificazione che non raggiunge il suo

è una semplificazione, e una semplicità che costano tanta fatica e che, qualche volta, sono più facili da realizzare quando una cultura, uno spirito e una storia forse aiutano. Bisognerebbe forse vedere il mondo dalla parte dei fragili. Questo

Signor Presidente, farò una dichiarazione di voto molto breve, perché penso di avere già utilizzato molto del nostro tempo illustrando la mozione che la Lega Nord ha presentato su questo argomento molto importante. Voglio soltanto mettere in In primo luogo, la direttiva europea attualmente in vigore sui prodotti dietetici

obese e in sovrappeso o malnutrite, nonché prodotti a fini medici speciali, alimenti per allergici e intolleranti, fra i quali anche i celiaci, e alimenti specifici per gli sportivi.

cancellando quindi quella speciale tutela per i consumatori vulnerabili che ha funzionato per oltre 35 anni. Questo è il primo elemento

da quando è entrato in vigore il nuovo trattato di Lisbona (1° dicembre 2009), all'unanimità un parere nettamente contrario, sia dal punto di vista del principio della proporzionalità che della sussidiarietà, oltre che del merito. Questo è il secondo concetto

È vero che è prioritaria la tutela della salute dei cittadini italiani ed europei, ma ricordo che l'industria dei prodotti dietetici vale in Europa 24 miliardi di euro e che in Italia muove un fatturato di 1,5 miliardi di euro l'anno, tra multinazionali e piccole e medie imprese. In Europa vengono investiti ogni anno 1,2 miliardi di euro in innovazione, ricerca e studi sulla produzione di questi alimenti particolari. Valori molto alti, che garantiscono la qualità e, quindi, la sicurezza per il consumatore e le categorie protette. Valori dunque molto alti - dicevo - rispetto ai settori dell'industria alimentare in generale, che verrebbero decisamente resi nulli e ridicolizzati da questa proposta di deregolamentazione avanzata dalla Commissione europea. Questo non è un passaggio da poco. È vero che prioritariamente bisogna garantire la

le mozioni presentano elementi peculiari e conducono alle stesse finalità: evitare che una legislazione nazionale, senza dubbio all'avanguardia, debba essere ridimensionata per far fronte all'esigenza di adeguarsi alla normativa europea. L'impegno richiesto al Governo è di far valere con ogni mezzo e strumento a disposizione le proprie ragioni che sono valide ed efficaci intanto perché garantiscono maggiore tutela ai malati di celiachia. Non si tratta qui di tutelare un prodotto o una prerogativa italiana, bensì di seguire procedure che devono in ogni modo evitare che ci possa essere confusione o comunque che si possano creare presupposti per l'aggiramento di norme che - lo ripeto - sono state emanate a tutela dei malati di celiachia.

E' materia troppo delicata e troppo diffusa, in particolare tra i bambini, per cui è necessario un intervento del Governo determinato ed intransigente. Come giustamente si esplicita nelle mozioni, la proposta COM 353 cancellerebbe, di fatto, dalle etichette dei prodotti alimentari la definizione «prodotto dietetico» riducendo la dicitura «senza glutine» ad un'etichetta molto generica. In definitiva, si è cercato di affrontare con una legislazione adeguata le problematiche dell'etichettatura in genere sui prodotti alimentari; immaginiamo come sarebbe devastante su prodotti destinati ai malati di celiachia,

Sappiamo che la celiachia è una malattia che ad oggi conosce come unica terapia l'astensione dal consumo di prodotti con glutine. In questi anni l'etichetta "prodotto dietetico senza glutine" è stato un importante obiettivo per quanti affetti da tale malattia. Grazie, infatti, a questa dicitura sono entrati nel mercato prodotti sempre più vari che permettono anche ai celiaci di perseguire una dieta variegata. Cancellando la definizione di "prodotto dietetico", si ridurrebbe la dicitura "senza glutine" ad un semplice *claim* da apporre in etichetta. Anche l'Associazione italiana celiachia, insieme ad altre associazioni europee, si sta mobilitando contro questo provvedimento in cui sono certi di vedere calpestati i diritti e le garanzie per la salute di tutti quei cittadini affetti da tale patologia. Il risultato sarebbe quello di ottenere due effetti gravi: la perdita delle garanzie legate alle regole fondamentali perché un prodotto possa essere considerato adatto per chi non deve consumare glutine; per quanto riguarda il nostro Paese, l'abrogazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (norma nazionale di recepimento delle direttive europee sui dietetici), e, come conseguenza, la cancellazione dal Registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine, strumento utile ai celiaci perché raccoglie i

Gruppo del PdL, attraverso il senatore D'Ambrosio Lettieri, si è mosso sin dal primo momento in modo energico per poter raggiungere tale risultato. Permettetemi di dichiarare l'apprezzamento per le parole pronunciate dal Ministro e la totale fiducia che il Governo farà tutto quanto è in suo potere per l'adozione in ambito europeo, e non solo,

L'abolizione della definizione di prodotti dietetici e la riduzione della dicitura senza glutine ad un'etichetta generica, con la proposta che diventino alimenti di consumo corrente, farebbero venir meno la protezione riservata ai celiaci, una tutela garantita da una stringente normativa sui requisiti nutrizionali specifici e sui controlli relativi. non si può, in nome della semplificazione e dell'armonizzazione legislativa, mettere a repentaglio la salute di una categoria di pazienti che ad oggi necessitano come unica terapia di una dieta alimentare priva di glutine. Stiamo parlando nella sola Italia di circa 80.000 pazienti e di 350.000 persone non ancora diagnosticate, secondo le ultime stime, che chiedono di vedere garantito il loro diritto a continuare ad usufruire, senza timore di alcun rischio, di cibo senza glutine. Le norme si cambiano per far crescere il progresso di una società e non certo per sancire una regressione nella tutela dei diritti dei cittadini più vulnerabili. Le norme attuali hanno funzionato. È innegabile che soltanto il regolamento CE, provvedimento tra l'altro recente e rispondente ai bisogni dei celiaci, insieme alle linee guida già trasmesse dal Ministero della salute, prevedendo che la dicitura «senza glutine» sui prodotti sia riportata soltanto dopo rigorose procedure e controlli, e controlli, sia l'unico strumento che tutela la salute stessa del celiaco che sa di poter nutrirsi senza rischi. Va inoltre ricordato che in Italia questi prodotti sono elencati nel Registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine ed erogati gratuitamente ai celiaci dal Sistema sanitario nazionale.

per i quali un accertamento rapido della patologia significa allungare loro la vita. Concludendo, come dichiarato in apertura, sono certo che il Governo si impegnerà a promuovere e a dare seguito alla mozione oggetto della nostra discussione. Non potrebbe essere diversamente considerando che, pochi giorni fa, in occasione del vertice delle Nazioni Unite sulla prevenzione e sul controllo delle malattie non trasmissibili, svoltosi a New York, il ministro Fazio ha ricordato che l'Italia ha già messo in campo il programma «Guadagnare salute», il quale annovera tra i suoi punti cardine l'importanza della sana alimentazione. Sarebbe davvero una contraddizione grave non proteggere i celiaci, che necessitano come unica terapia di una sana alimentazione priva di glutine. finestra"). Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Signor Presidente, sottosegretario Gioachino, onorevoli colleghi, colleghi, con la presentazione di questa mozione abbiamo inteso gettare uno squarcio di luce sulla situazione di crisi che da tempo investe il settore dell'autotrasporto nel nostro Paese, consapevoli che ben altri e più rilevanti riflettori sono necessari per fare piena luce su questo delicato e strategico comparto. Le questioni che con la nostra mozione vengono poste in evidenza sono, come tutti tutti i punti di osservazione, di per sé parziali e non esaustive di una realtà tanto complessa e contraddittoria, che come tale va analizzata, giudicata e, se ci riusciamo, orientata e corretta. Molteplici ed evidenti distorsioni nella regolazione di questo settore ci inducono ad un severo giudizio nei confronti dell'azione di Governo di questi anni. Proprio per questo intendiamo sfidare il Governo, indicando politiche e azioni, da noi ritenute essenziali, che vogliamo sottoporre, alla luce del sole e nelle più autorevoli sedi istituzionali, all'attenzione del Paese e dei diretti interessati, e sulle quali vi invitiamo fin da ora a pronunciarvi e a rendere conto. Partiamo da pochi ma essenziali dati: il settore dell'autotrasporto in Italia vanta più di 90.000 imprese, il doppio di quelle in Francia (poco meno di 45.000) e il triplo di quelle in Germania (poco più di 30.000). Il settore dell'autotrasporto nel nostro Paese è il comparto del trasporto merci più assistito dalle politiche pubbliche (circa 5 miliardi di euro solo negli ultimi sette anni),

Abbiamo volutamente selezionato questi aspetti, più di altri che avremmo potuto enumerare, perché a nostro avviso sono paradigmatici di una situazione paradossale che il settore dell'autotrasporto sconta nel nostro Paese. Si tratta di dati che meritano pertanto un loro disvelamento, per un'urgente correzione di rotta. Partiamo con i dati dimensionali. Alle quasi 100.000 imprese esistenti se ne aggiungono in realtà altre 50.000 fittizie, imprese che non detengono materialmente la ragione sociale della loro attività: tradotto volgarmente, aziende che non hanno dotazione patrimoniale, neppure la motrice che serve loro per l'attività, talvolta, neppure dipendenti. Sono quindi imprese, nel migliore dei casi, di meri prestatori di manodopera, che allungano con la loro intermediazione la catena dei subappalti, o talvolta, si tratta di semplici scatole vuote. Anche le non trascurabili sovvenzioni che il settore riceve meritano una qualche precisazione: 4,9 miliardi di euro negli ultimi sette anni; oltre 700 milioni solo nell'ultimo anno, erogati sotto forma di sconti sulle accise ai carburanti, piuttosto che alle polizze assicurative o alla riduzione dei pedaggi autostradali. Sono per lo più risorse che il mondo dell'autotrasporto vede in minima parte e che quasi mai vanno nelle tasche degli autotrasportatori, ma che invece alimentano surrettiziamente gli stessi petrolieri, le assicurazioni e i concessionari autostradali; sembrerà strano, ma proprio quei signori che il Ministro dell'economia aveva dichiarato di mettere sotto torchio e che non a caso - dico io - ridevano di quelle improvvide dichiarazioni. Infine, i dati sulla sicurezza stradale, a dir poco eloquenti. I progressi fatti dalla legislazione e dalle azioni di prevenzione, sia con i Governi di centrodestra che con quelli di centrosinistra, in perfetto stile *bipartisan* (come si usa dire), sono stati considerevoli. Eppure, se c'è un settore che arretra è proprio quello dell'autotrasporto, e stiamo parlando di indiscussi professionisti della strada. Evidentemente qualcosa stride nei controlli che non verificano le effettive condizioni di lavoro. Questi tre macrodati evidenziano un settore ipertrofico e frammentato, ma anche estremamente fragile per quanto strategico ed essenziale all'economia del Paese. Sappiamo tutti, senza evocare questa volta scenari cileni fuori luogo, vista anche la penetrazione della criminalità organizzata nel settore, che un blocco del comparto per più giorni metterebbe in ginocchio il Paese e produrrebbe danni economici incalcolabili. Un settore che ciò nonostante è caratterizzato da una concorrenza asimmetrica tra gli stessi operatori del settore, perché le regole non sono, come è evidente, uguali per tutti, e dove la competizione, fatta essenzialmente sui costi, è soggetta a controlli limitati e sanzioni discutibili, quando vengono applicate. Da qui la preoccupazione da parte nostra che state maneggiando incautamente "roba" assai pericolosa. Dal punto di vista della politica industriale del comparto, si sono generati negli anni ulteriori paradossi e distorsioni di sistema che voglio passare rapidamente in rassegna. Nonostante gli incentivi erogati, le imprese sono rimaste per fatturato, addetti e investimenti ferme a come erano nel 2000. Si è favorita una competizione disumana delle regole del mercato, in quanto essenzialmente orientata ad una compressione dei costi a scapito di sicurezza e qualità ambientale, facendo venire meno il principio comunitario di «chi inquina paga», ma anche consentendo l'interpretazione di una politica di delocalizzazione sconsiderata, sfruttando irregolarmente la libertà di stabilimento attraverso la finta apertura di sedi all'estero. Il risultato più clamoroso è che le imprese più strutturate sono anche quelle più a rischio. un settore privo di una politica industriale degna di un Paese che si ostina a definirsi avanzato. Verrebbe da dire, in evidente polemica, che l'autotrasporto costituisce solo una ulteriore variante dei singolari processi di liberalizzazione che il settore dei trasporti in questo Paese ha conosciuto. Liberalizzazioni che hanno finito per essere tutto, meno che ambiti regolati in cui la concorrenza si sviluppa in sicurezza, secondo standard predefiniti, validi per tutti gli operatori e sulla qualità del servizio erogato. Chi ne ha fatto le spese sono stati soprattutto i lavoratori, costretti a condizioni di lavoro proibitive, fuori, troppo spesso, dagli ambiti apparenti della legalità formale. Ripeto, stiamo parlando di un settore strategico per la filiera dell'industria nel trasporto delle merci, soprattutto per la flessibilità che garantisce nel servizio. È però l'anello più debole della catena logistica del Paese e, come per ogni catena, è proprio dagli anelli più deboli che si misura la forza del sistema. Rafforzarlo significa rafforzare l'intero sistema e per farlo occorre perseguire alcune strategie di fondo essenziali. si chiama integrazione modale e significa superare la contrapposizione storica gomma - rotaia determinando invece le convenienze di incontro per entrambi i settori con politiche di incentivi allo scopo finalizzati, a partire da quelli che erano stati previsti per l'incremento delle autostrade del mare, che voi avete invece scelleratamente definanziato e che costituivano un obiettivo strategico, proprio per un Paese dalle non agevoli caratteristiche orografiche come il nostro. La seconda consiste nel favorire una politica industriale vera del settore, offrendo una visione di sistema e agevolando la formazione di imprese di trasporto di dimensioni industriali, superandone l'attuale frammentazione, con incentivi volti a favorirne l'aggregazione. La terza strategia presuppone una politica logistica nel nostro Paese attualmente inesistente, e su cui però si gioca la vera sfida di competizione nella distribuzione dei prodotti, in entrata e in uscita, sia dal Paese che dalle realtà urbane e metropolitane, superando il congestionamento e lo stazionamento delle merci. Per realizzare tutto ciò occorre una ristrutturazione del comparto e una riorganizzazione del servizio in grado di assorbire i maggiori costi determinati da quelle che in gergo si chiamano le rotture di carico. Rendere conveniente anziché costoso il trasferimento delle merci da un vettore all'altro all'altro è possibile solo con grandi soggetti industriali e con la previsione di processi di lavorazione aggiuntivi ad ogni rottura di carico, appunto. Per fare ciò occorre rimuovere tutti i principali fattori che ostacolano questo processo e disincentivare ogni forma di intermediazione

incentivare l'acquisizione delle imprese che chiudono, favorendone l'acquisizione da parte di altre imprese italiane, garantendo sgravi fiscali e contributivi a coloro che ne assumono il personale e i mezzi; prevedere la confisca della merce in caso di trasporto abusivo e mancato rispetto della normativa in materia di costi minimi; assumere iniziative atte a contenere il fenomeno della subvezione, limitando a due passaggi la vendita dello stesso contratto di trasporto; inasprire il sistema dei controlli nei confronti delle imprese che violano il codice della strada e delle imprese che sfruttano irregolarmente la libertà di stabilimento attraverso la finta apertura di sedi all'estero; prevedere nuove norme per impedire, indipendentemente dalla natura sociale dell'impresa, le violazioni in termini di sicurezza o di tutela delle condizioni di lavoro dell'autotrasportatore. Ecco, Ecco, Sottosegretario, siamo consapevoli che queste non sono riforme a costo zero, come quelle elencate nel piano della logistica - a lei caro - ma che purtroppo non saranno fatte proprio perché, essendo apparentemente a costo zero, hanno un costo maggiore di queste, andando a mettere in discussione dieci anni fa al Paese e che non avete realizzato. Questi invece sono provvedimenti da fare subito, che costano probabilmente meno delle sovvenzioni che annualmente vengono apparentemente erogate al settore e che guardano al futuro del Paese. Quello che vi chiediamo è di farci capire e far capire agli italiani se questo Paese lo volete governare, rischiando, inevitabilmente nella situazione data, un po' del vostro residuale consenso, o se pensate solo alla vostra improbabile sopravvivenza. Purtroppo per il Paese, come è ormai ben chiaro, la questione che vi poniamo, non riguarda solo l'autotrasporto. Signor Presidente, colleghi senatori, signor Sottosegretario, come ricorderà bene il sottosegretario Giachino, in quanto ha partecipato al convegno tenutosi a marzo 2011 sull'autotrasporto, l'Italia dei Valori si è interessata particolarmente a questo tema, perché siamo convinti dell'importanza del settore per la nostra economia e riteniamo che l'autotrasporto sia una componente fondamentale della catena logistica, soprattutto in un Paese in cui, volente o nolente, le merci vengono spostate principalmente ancora su gomma. Ma siamo anche convinti che le politiche sinora poste in essere in materia, in particolare negli ultimi dieci anni, non abbiano conseguito gli effetti sperati di effettivo sostegno al settore, per garantire allo stesso autonomia e competitività. Da più di dieci anni a questa parte, lo Stato paga cifre esorbitanti per sostenere il settore dell'autotrasporto. Solo nel decennio 2000-2009 sono stati spesi 3,5 miliardi di euro in favore dell'autotrasporto con una serie, però, di interventi a pioggia - qui sta il problema - che troppo spesso hanno avuto carattere di pura assistenza. Non sono stati finalizzati e soprattutto, a nostro avviso, non sono andati a beneficio del rilancio del settore. Troppo spesso dell'autotrasporto ci si ricorda in campagna elettorale o quando la categoria risente di particolari problemi - come sta accadendo in questo periodo - magari minacciando un fermo con conseguenze economiche importanti. È mancata una vera politica che fosse espressione di una visione d'insieme, di una volontà di autentica riforma della disciplina. Questo ha fatto sì che il sistema rimanesse frammentato, polverizzato, con un numero di imprese che è andato aumentando, comportando una netta perdita di competitività del settore soprattutto in termini di organizzazione ed innovazione tecnologica ed esponendo i nostri vettori, in particolar modo i padroncini, alla concorrenza, spesso sleale, dei Paesi dell'Est. Il settore è dunque in sofferenza per i costi del lavoro (più elevati in Italia rispetto ad altri Paesi) e per i costi del carburante che sicuramente hanno un'incidenza notevole nel conto economico di un'impresa. Quello che noi diciamo è che le risorse vanno assegnate come accompagnamento alle imprese, come chiediamo per tutti i settori, soprattutto in un momento critico come quello attuale, ma vanno riorganizzate e assegnate secondo altre logiche. logiche. Voglio dire che bisogna smetterla di fare ricorso alla logica del sussidio e soprattutto di difendere inefficienze strutturali con misure orientate al ritorno a sistemi paratariffari e anticoncorrenziali. Non siamo d'accordo senza dubbio sul modo di legiferare adottato per intervenire in questo settore. Non posso dimenticare che avete inserito in un decreto-legge vertente su tutt'altra materia i contenuti di un protocollo d'intesa concluso sotto la minaccia di un fermo dei servizi, con il dissenso della committenza e il parere contrario dell'*Antitrust*. Siamo convinti invece che ci sia bisogno di ampio confronto, che sia giunto il momento di definire un quadro di riferimento all'interno del quale si possano individuare finalità, priorità e risorse per il rilancio del settore, con precisi impegni dello Stato al fine di orientare le strategie dei diversi soggetti imprenditoriali coinvolti. Riteniamo necessario addivenire quanto prima ad una riforma organica della disciplina del settore dell'autotrasporto, nel pieno rispetto dei principi della concorrenza, della trasparenza, della tutela della sicurezza stradale e della sicurezza sul mezzo di trasporto. Quello che noi proponiamo al Governo è di procedere ad una definitiva liberalizzazione del mercato attraverso il superamento dell'attuale meccanismo dei costi minimi di esercizio, prevedendo una clausola di legge di eccessiva onerosità sopravvenuta per il contratto di trasporto che sia in grado di salvaguardare la posizione giuridica di entrambi i contraenti nel momento in cui si verifichino oscillazioni rilevanti dei prezzi degli idrocarburi, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Vi è poi un fenomeno importante che vi chiediamo di affrontare immediatamente: la cancellazione immediata dagli albi provinciali delle 50.000 imprese prive di veicoli. impedisce di creare reali condizioni di trasparenza sul fronte dell'offerta. Tali aziende infatti, dette anche agenzie cosiddette intermediarie di autotrasporto, operano senza avere veicoli, ma acquisiscono commesse e le girano ad altre imprese a prezzi ovviamente più bassi, alimentando una lunghissima catena di subappalti che poi finisce per strozzare il vettore effettivo che deve eseguire il trasporto. Verrebbe da chiedersi perché succede tutto questo e la risposta è molto semplice: innanzitutto perché per iscriversi all'albo occorre dichiarare il possesso di almeno un veicolo, ma nei fatti il veicolo stesso può essere venduto anche il giorno dopo la sua registrazione. Mi chiedo se non avrebbe senso, a questo punto, valutare una modifica del decreto legislativo n. 112 del 1998 per togliere la competenza alle Province in materia di tenuta degli albi. L'Italia dei Valori propone da tempo la soppressione delle Province che, neanche a farlo apposta, pure nel settore dell'autotrasporto, hanno solo contribuito a generare confusione e dispendio di tempo e risorse. Analogamente, riteniamo vada affrontato il tema dell'incentivazione per favorire le aggregazioni e le fusioni tra imprese di autotrasporto. In Italia quasi la metà è proprietaria di un solo veicolo ed oltre la metà delle imprese è costituita ancora da ditte individuali. Questo dato rende difficile la sopravvivenza delle stesse imprese sul mercato. Ci sono stati interventi per favorire l'aggregazione. Ricordo per tutti che nel 1997 l'allora ministro Burlando tentò di perseguire la strada degli incentivi per l'aggregazione, ma a distanza di anni è evidente che quella strategia non ha funzionato. Ad avviso dell'Italia dei Valori, questi incentivi dovrebbero essere concessi in modo proporzionale all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a seguito dell'operazione di aggregazione o di fusione e, soprattutto, in relazione al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa prima della conclusione dell'operazione di aggregazione o di fusione, purché il numero finale dei veicoli, una volta conclusasi la predetta operazione, non risulti inferiore alle 10 unità. Gli incentivi potrebbero essere concessi sotto forma di sgravi fiscali e contributivi legati all'incremento della base occupazionale. L'obiettivo deve essere quello di assegnare le risorse con la precisa finalità di giungere all'aggregazione e non come è accaduto con il cosiddetto milleproproghe di attribuire genericamente ben 246 milioni di euro ad interventi di sostegno del settore dell'autotrasporto, senza specificare in concreto la finalità. Altro punto per noi fondamentale è quello dell'innovazione tecnologica. E sappiamo che innovare costa alle imprese. Riteniamo necessario supportare questi investimenti. C'è poi il problema della responsabilità del vettore. Tale intervento riguarda il limite del risarcimento. La prassi ha dimostrato che il limite allora pensato a favore dei vettori è risultato un *boomerang*, in quanto a seguito della sua introduzione vi è stato un aumento del contenzioso volto a superare tale limite adducendo la colpa grave del vettore, con importanti riflessi anche assicurativi. Noi crediamo che prevedere un limite sensibilmente più alto di quello previsto dalla normativa interna, uniformandolo a quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra, così come ha fatto la Germania, garantirebbe una maggiore adeguatezza dei risarcimenti ed un maggior grado di certezza. Ultimo punto, ma ovviamente non meno importante, quello dei controlli e della concorrenza sleale. Vi è un numero sempre crescente di veicoli industriali provenienti dai Paesi nuovi entranti nell'Unione europea, che operano nella più totale mancanza di rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, a causa di un'assenza di regole certe e di una scarsa politica dei controlli a livello europeo e nazionale. Questo comporta una situazione drammatica per l'autotrasporto italiano e per l'economia ad esso collegata. Per tali ragioni, l'Italia dei Valori ritiene prioritario che il Governo si adoperi presso le competenti istituzioni comunitarie al fine di giungere all'adozione di una serie di misure *antidumping.* In ambito nazionale riteniamo poi importante che venga garantita la necessità di uniformare i controlli su tutto il territorio nazionale, sia quelli di tipo fiscale e previdenziale che quelli in materia di sicurezza dei mezzi di trasporto circolanti. Concludo dicendo che i temi che riguardano il settore e che andrebbero affrontati sono certamente diversi e molteplici. C'è il problema dell'ecosostenibilità e dell'intermodalità, per noi fondamentali; quello dei viaggi a vuoto; dei ferrobonus, ed altri ancora, ma auspichiamo che intanto, onorevole sottosegretario Giachino, si possa trovare condivisione sulla necessita di procedere con un approccio integrato di sistema, in grado di garantire la crescita della competitività del nostro autotrasporto, smettendola con la strategia degli interventi a pioggia o di carattere emergenziale.

ha illustrato con dovizia di particolari le motivazioni che, a nostro parere, rendono questa mozione una proposta molto seria cui sarebbe opportuno che maggioranza e Governo dessero ascolto e seguito. Mi limiterò quindi a qualche considerazione sulle criticità del settore e sulla necessità di superare ed archiviare definitivamente la politica degli incentivi a pioggia per passare ad una politica fatta, sì, anche di incentivi, ma di incentivi dati in cambio di regole e del loro rispetto. Infatti, signor Sottosegretario, come ha brevemente ricordato il senatore Marco Filippi, circa un anno fa, nel rispondere proprio ad un mio intervento critico sulle generose provvidenze del Governo a favore dell'autotrasporto, nel difendere le iniziative dell'Esecutivo, sostenne che grazie ad esse si era scongiurato il pericolo di agitazioni e scioperi nel settore. Trascinato evidentemente dall'entusiasmo e dalla foga, giunse addirittura a sostenere che si era scongiurata la paralisi del Paese e, non contento, mi invitò a non dimenticare quanto nei primi anni Settanta era successo nel Cile di Allende sulla deriva degli scioperi dell'autotrasporto. In buona sostanza, il messaggio del Governo si poteva sintetizzare così: non si può scherzare con questo settore perché, se si ferma il trasporto su gomma, si ferma il Paese. Complimenti, in primo luogo, per la schiena diritta. In secondo luogo, per la lungimiranza politica: invece di mettere mano al sistema, dandogli sì misure di sostegno ma anche e soprattutto regole, si preferisce evidentemente la linea delle concessioni e degli incentivi senza chiedere nulla in cambio se non una labile garanzia di pace sociale. Centotrentaquattro milioni di euro di riduzione di premio INAIL; 174 per la detrazione forfetaria di spese non documentate; 54 per la riduzione della tassa di possesso; 15 per il fondo d'investimento; 77 per l'ecobonus; 50 per il Fondo di garanzia delle piccole e medie industrie; 137 di riduzione dei pedaggi autostradali: questo è solo un breve ed incompleto elenco degli incentivi decisi nel 2009 a favore degli autotrasportatori e sostanzialmente interamente confermati nel 2010 e nel 2011. Peccato che questo fiume, o questi fiumiciattoli, di denaro non abbiano inciso minimamente sulla struttura di impresa né sulla qualità delle imprese che vivono ancora e nuovamente oggi una situazione drammatica. Se si guarda poi alla struttura delle voci di spesa di queste imprese, si vede come si tratti di voci non comprimibili (parliamo di carburanti, di costo dei mezzi e via dicendo),

come è stato detto prima, composto da 90.000 aziende che gestiscono mezzi e conducenti che ogni giorno effettuano spostamenti più o meno lunghi sulle strade nazionali ed internazionali. La morfologia del nostro territorio e la carenza di infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie contribuiscono a fare dell'autotrasporto un'attività sicuramente di primaria importanza per l'intera economia nazionale. Il comparto è in crisi - lo sappiamo - e si deve scongiurare la chiusura delle imprese e l'alterazione del regolare servizio di movimentazione delle merci, che rappresenta per il nostro sistema produttivo, per la grande distribuzione e, quindi, per l'intera collettività una risorsa primaria. Ecco perché il Governo è intervenuto massicciamente in questo settore negli ultimi 40 mesi, cercando di difenderlo al meglio dalla crisi con l'aumento di 200 milioni l'anno e lavorando con il nuovo Piano nazionale della logistica, proprio per rendere più competitiva la logistica italiana, per farle acquisire nuovi traffici e quindi nuova domanda di trasporto, potenziando i servizi di trasporto e di logistica, per promuovere l'adozione di modelli logistici ottimali per filiere specifiche, per incoraggiare lo sviluppo di standard operativi fondati su forme di aggregazione peculiari del settore.

nostro Paese, stimata in circa 40 miliardi di euro annui, attraverso dieci linee strategiche e 51 azioni che interessano i diversi settori dei trasporti e della logistica, nonché le norme, le regole e la valutazione degli effetti degli interventi che saranno realizzati. Nel corso del 2011, la Consulta ha portato avanti le linee di attuazione del Piano, dando vita ad approfondimenti tematici nel campo dell'intermodalità ferroviaria e marittima, sulle piattaforme territoriali e sui principali processi di filiera di filiera (agroalimentare, la distribuzione urbana delle merci, *reverse logistics*, merci pericolose, farmaco), con l'obiettivo di abbattere i costi logistici, diffondere le tecnologie ITS (*Intelligence Transport System*), ridurre i tempi di attraversamento dei porti e razionalizzare le operazioni di carico e di scarico. Entro quest'anno è previsto che vengano avviate le sperimentazioni, finanziate dalla Consulta, previste da accordi con le istituzioni e le associazioni interessate. Non dimentichiamo mai che all'autotrasporto italiano si sono dedicate negli ultimi vent'anni personalità politiche di rilievo, da Bernini, a Burlando, a Bersani Treu. Lascio a chi conosce il settore la valutazione di quello che è stato fatto in questi vent'anni da queste persone, malgrado i notevoli incentivi che sono stati dedicati al comparto. Sicuramente il settore dell'autotrasporto risente di una serie di squilibri e di carenze strutturali che, unitamente alla congiuntura economica sfavorevole, minano la competitività delle nostre imprese a vantaggio di quelle straniere, come è stato già ricordato. Il percorso Il percorso di liberalizzazione regolata, intrapreso in questi anni, deve essere portato avanti, con l'obiettivo di migliorare la mobilità delle merci e di renderla competitiva nel contesto europeo. Per quanto riguarda l'attività di controllo in questi ultimi anni, mi risulta che la Polizia stradale effettui regolarmente controlli sui camion e i mezzi pesanti che circolano sulle strade, per verificare il rispetto, da parte dei vettori nazionali, comunitari ed extracomunitari, delle disposizioni vigenti in materia di tempi di guida, pause e riposi degli autisti, e delle altre disposizioni volte a garantire la sicurezza sulle nostre strade. Mi sembra doveroso puntare a favorire, anche attraverso una forte e rinnovata politica dei controlli, comportamenti rispettosi delle norme a tutela della concorrenza, e, contestualmente, puntare a politiche che rendano

i dati contenuti nel rapporto biennale della Commissione europea sui controlli relativi al periodo 2007-2008 da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Le verifiche sul rispetto del regolamento comunitario sui tempi di guida e di riposo evidenziano che gli accertamenti sono stati effettuati, nell'80 per cento su veicoli e autisti nazionali, mentre in altri Paesi la tendenza è invertita e i controlli sono stati effettuati per la maggior parte sui veicoli stranieri. Sicuramente una politica di controlli congiunti fra l'Italia e i Paesi confinanti potrebbe essere più fruttuosa e produttiva per sviluppare una cooperazione operativa, che porti ad elevare gli standard di sicurezza stradale e, contemporaneamente, a combattere la concorrenza sleale.

Così come sarebbe opportuno distribuire in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale le attività ispettive, non concentrandole solamente su alcune aree, ciò che comporta una evidente penalizzazione per chi opera in quei territori. È anche necessario intervenire per superare le abitudini commerciali degli operatori italiani nelle transazioni con l'estero. Considerata anche la forte vocazione esportatrice dell'Italia, il fatto che la regia dell'attività di logistica sia lasciata agli operatori esteri rappresenta una perdita di fatturato, stimata nell'ordine di 10 miliardi di euro l'anno, che il nostro sistema economico non può più permettersi. Per affrontare le diverse criticità sollevate dagli operatori del settore e per rilanciare l'intero sistema, il Governo ha quindi ritenuto importante costituire un Tavolo permanente Una condivisione di obiettivi tra la committenza ed il comparto può essere il punto essenziale da cui ripartire per definire una piattaforma comune verso un sistema di trasporto competitivo, regolare e sicuro. Grazie al lavoro di questo tavolo sono state introdotte regole volte a favorire la trasparenza del mercato ed una maggiore correttezza nei rapporti fra la committenza e gli autotrasportatori: costi minimi di sicurezza anche per i contratti scritti, da individuare nell'ambito di accordi di settore; tempi di pagamento non superiori a 60 giorni dall'emissione della fattura per i servizi di trasporto; disciplina dei tempi di carico e scarico; possibilità di azione diretta da parte di chi esegue effettivamente il trasporto nei confronti del committente originario,

globale in atto: il nostro autotrasporto, infatti, è probabilmente uno dei comparti economici più colpiti dalla crisi, tanto che questa maggioranza ha

Ma il metodo del confronto fra le parti interessate, la condivisione e lo spirito propositivo penso che siano il modo migliore per risollevare l'intero sistema.

alla distribuzione urbana delle merci e alla ricerca di un miglior equilibrio commerciale tra vettori e committenza, per una crescita della capacità competitiva delle imprese. Un aspetto importante sono gli interventi di ordine burocratico, come la previsione di una deroga per l'esame di idoneità professionale per le aziende che hanno alle spalle anni di attività regolare senza rilievi, che potrebbero dare un po' di respiro agli autotrasportatori. in alcune province la percentuale dei non idonei è altissima, anche perché non è pensabile che un titolare di licenza, in questo delicato periodo economico, tralasci il lavoro per dedicarsi completamente allo studio. affinare ed individuare nuove aree di convergenza e di crescita complessiva del sistema trasportistico nazionale debba essere alla base dell'intero lavoro per raggiungere il risultato virtuoso di una maggiore trasparenza, efficienza e crescita nel settore dell'autotrasporto.

la proposta che noi avanziamo parte, tra le varie cose, anche da una considerazione che deriva da una semplice analisi di politica industriale:

Germania. Cosa c'entra questa comparazione dei dati? C'entra, perché il settore dell'autotrasporto è l'elemento di maggiore inefficienza del nostro sistema economico. Da un lato, si è concentrata la logistica, soprattutto dal punto di vista finanziario, dall'altro si è concentrata, o almeno in parte sta concentrandosi, l'industria, cioè la committenza. Tutti sappiamo che per stare sulla scala della competizione globale sono necessari fenomeni di concentrazione e nel contempo Ciò che mette in relazione mercati e produttori è l'autotrasporto e questo non si è concentrato, è rimasto fortemente polverizzato, con una condizione di vita dell'autotrasportatore italiano che credo sia paragonabile soltanto a quella dei raccoglitori di frutta nel Mezzogiorno, quando vengono chiamati abusivamente a raccogliere la frutta e a lavorare in nero.

personale e imprenditoriale e quella delle loro famiglie al debito che hanno contratto per tutta la vita. Si sono trasferiti, come si è detto qua, molti soldi all'autotrasporto.

Sono in realtà soldi che sono serviti a comprimere ulteriormente i costi del servizio di autotrasporto per il committente e il destinatario. Si sono compressi i prezzi e si sono pagati molti soldi pubblici; il mercato è stato violato ancora una volta e la competizione non ha vinto: ha vinto un costo pubblico che ha consentito a petrolieri e a committenti di varia natura di accrescere le proprie ricchezze, non sul piano competitivo ma sul piano dello sfruttamento di un segmento della catena di costruzione del valore. Non abbiamo mai valorizzato l'autotrasporto come una componente della catena di costruzione del valore del prodotto, e quindi siamo un Paese più debole. Siamo un Paese che non fa intermodalità perché non investe sul trasporto ferroviario; siamo un Paese più debole perché ha preferito avere una miriade di debolissimi autotrasportatori piuttosto che finalizzare una parte di quegli incentivi all'aggregazione tra imprese, alla nascita di imprese più strutturate

Mi capitava proprio l'altro giorno di incontrare soci di una società di persone del settore dell'autotrasporto i quali, per attrarre capitali, avevano intenzione di trasformarsi in società di capitali. All'albo dell'autotrasporto questo vuol dire bloccare la propria attività dai tre ai sei mesi, perché il mero cambio societario blocca l'attività di queste imprese. imprese. Non è un grande costo fare in modo che una società di persone, diventando società a responsabilità limitata o crescendo nella sua struttura societaria, possa immediatamente continuare la propria attività,

Che non la si voglia è evidente non tanto dalla quantità di denaro che viene speso e sulla quale tutti i diversi *stakeholder* guadagnano moltissimo (dalle autostrade, ai rivenditori di carburanti, a quelli che hanno il prezzo dell'autotrasporto più basso d'Europa, ma anche il servizio più inefficiente d'Europa), lo stretto rapporto che c'è tra funzionamento dell'autotrasporto e funzionamento del sistema industriale del nostro Paese. Forse quei numeri ci dicono qualcosa di più: di più: che siamo poco competitivi perché abbiamo preferito tenere non un sistema di piccole imprese, ma una miriade di disperati. Le piccole imprese sono un'altra cosa: sono forme che si organizzano tra loro

non della grande impresa, ma dell'impresa grande, cioè delle imprese piccole che si aggregano tra di loro per fare produzione lavoro, trovare nuovi mercati, avere nuovi strumenti di collegamento, per poter partire da Milano per fare un carico ad Instanbul e trovare qualcuno di fianco ad Instanbul

il quale, però, garantisce un prezzo più basso delle flotte di quei Paesi. Lo fa solo sulla propria pelle e pagando un prezzo inaudito allo Stato e a un mercato che non è competitivo. Purtroppo, negli anni, il timore

è mai stata la volontà di fare una seria programmazione per modificare e riformare questo settore. Si minaccia un fermo; si stanziano dei quattrini per tacitarlo e non non ci si cura di sapere dove andranno. Mentre si minaccia un fermo e molta committenza protesta, la stessa sa che da quella minaccia e da quelll'impegno pubblico trarrà vantaggi ulteriori che non trarranno i trasportatori, con buona pace di questo settore, di questo mercato e della produttività del sistema Italia. Forse è arrivato il momento di trattare il trasporto come una parte fondamentale della politica industriale del nostro Paese.

anche di questioni che riguardano la crisi economica e finanziaria; qualche volta ci siamo impegnati a dire che non c'è c'era crisi economica e finanziaria, ma mai ci siamo impegnati a parlare neanche un briciolo di politica industriale. Mai abbiamo affrontato il tema della competitività del nostro Paese rispetto agli altri Paesi, e ci meravigliamo che non ci siano provvedimenti per la crescita, ma solo per il contenimento dei costi. Abbiamo abolito la politica energetica: non abbiamo abolito il nucleare, ma abbiamo abolito ogni politica energetica, perché avevamo puntato sull'energia nucleare per la nuova politica industriale e, saltata quella, non c'è un briciolo di idea alternativa. Non abbiamo alcuna idea per strutturare le nostre imprese nella competitività. Non agiamo su un settore di una delicatezza clamorosa come quello del trasporto, che è un settore che ha la stessa importanza nell'ambito delle capacità competitive del Paese, hanno la finanza, il settore delle comunicazioni, quello del trasferimento tecnologico e della ricerca. Siamo un Paese che vorrebbe stare nella competizione globale e che dovrebbe crescere. Abbiamo un sistema trasportistico che è certamente peggiore di quello dei più arretrati Paesi africani. Lo teniamo in questa condizione perché, come sempre, c'è qualcuno che, dal non avere una politica, ci guadagna. In Italia è sicuro che, dal non avere un mercato, tutti i monopolisti guadagnano e hanno sempre guadagnato: siano essi monopolisti

si dà qualche briciola per sopravvivere in una condizione di totale precarietà, senza concedere nulla che li faccia diventare imprese che stanno sul mercato competitivo.

Sottosegretario, con questa mozione noi mettiamo al centro, non la necessità di trasferire meno quattrini al settore dell'autotrasporto, ma di fare investimenti nel settore dell'autotrasporto. Non quattrini, ma investimenti per il futuro: credo che questa sia una soluzione sulla quale potremmo convergere, prima della prossima minaccia di fermo dell'autotrasporto.

perché mi piacerebbe molto convergere, a valle di una discussione come quella di oggi, sul tema autotrasporto, che un tema di grande delicatezza per l'importanza che questo sistema ha nel nostro Paese, visto che, comunque, oltre l'80 per cento delle merci vengono trasportate attraverso questo segmento industriale.

Io ricordo gli episodi più rilevanti, e poi entrerò nel merito, chiedendo al senatore Marco Filippi e ai cofirmatari della mozione di apportare alcuni correttivi per renderla compatibile con le nostre interpretazioni della crisi del settore. Premesso che parliamo di un settore cosiddetto industrialmente maturo, dove le condizioni di mercato subiscono soltanto in minima parte gli effetti dell'innovazione tecnologica, dell'organizzazione, eccetera (e quindi soggetto più di altri settori a fenomeni di *dumping*), malgrado questo, noi, nel 2005, facemmo un atto di coraggio promuovendo una legge di liberalizzazione del settore

che aveva come presupposto e come condizione per il suo funzionamento non soltanto il corretto comportamento degli attori della filiera, per i quali fu prevista una corresponsabilità nel caso del malfunzionamento dell'intera filiera:

Che cosa è accaduto sostanzialmente? La legge ha funzionato, tant'è che non si è più sentita l'esigenza di ritornare alle cosiddette tariffe a forcella, che sono state, dopo decenni, definitivamente abbandonate. E ha funzionato secondo me - perché dobbiamo vedere i problemi, ma dobbiamo cercare di dirci qualche volta in quest'Aula anche dove troviamo i bicchieri mezzi pieni, e non soltanto quelli mezzi vuoti sappiamo, i controlli (ce lo siamo detti tante volte in Commissione) sono fortemente aumentati ed è migliorato fortissimamente il panorama dei controlli.

i comportamenti individuali, quindi la necessità che i guidatori professionali, gli autotrasportatori, fossero totalmente esenti da rischi derivanti dall'uso penalizzammo ulteriormente comportamenti che non tenevano conto dei tempi di guida e di riposo. quindi un'ulteriore azione che andava nella direzione di favorire il processo di liberalizzazione con un quadro di controlli, da un lato, e un impianto normativo, dall'altro, sempre più adeguati.

e di comportamenti anomali che persistevano, stante la crisi finanziaria che già nel 2008 si era affacciata (una crisi finanziaria diventata poi anche crisi del manifatturiero, quindi una crisi industriale che è andata a incidere anche su un settore sensibile e vitale come l'autotrasporto), una cautela sui costi minimi del trasporto. È stato ed è un intervento estremamente rilevante, perché è a garanzia di questo sistema industriale che il mercato non arrivi ad alterare le condizioni minime di sicurezza, che sono ritenute un valore da apprezzare in modo assoluto e, quindi, da tutelare.

punti. Pur condividendo alcuni aspetti, mi lasciano tuttavia perplesso alcuni passaggi della mozione, che non condivido proprio in linea di principio.

di governo del settore, quasi come se da una cabina di regia centrale si riuscisse a disporre accorpamenti, fusioni e quant'altro: ciò è l'esatto contrario delle scelte operate dal Governo in tema di liberalizzazione e regolazione diversa del mercato.

l'incentivazione delle imprese che chiudono, con le «nuove disposizioni per le cooperative che impiegano soci lavoratori» l'assunzione «di iniziative per contenere il fenomeno della subvezione», eccetera. Quest'ultima richiesta è un'ulteriore criminalizzazione dei rapporti fiduciari. sia uno degli errori storici che hanno concorso a distruggere rami industriali del nostro Paese.

della qualificazione del rapporto, non è altro che una modalità di ampliamento della forza dell'impresa. Si tratta della modalità con cui un sistema come il nostro,

Questo è il sistema attraverso cui un'impresa si allarga e si impianta. Pertanto, dobbiamo stare attentissimi a toccare questi elementi, che sono importanti anche dal punto di vista finanziario. Mi spiego meglio: quando si fa ricorso a queste forme e ci si ritrova in difficoltà, tutto l'insieme risponde finanziariamente come se fosse un tutt'uno.

Signora Presidente, onorevoli senatori, le mozioni, anche se molto diverse, presentate dagli illustri senatori dell'opposizione, consentono di fare il punto nell'Aula parlamentare su un settore fondamentale per la nostra economia: l'autotrasporto. Circa il 90 per cento delle merci e dei servizi del nostro Paese, per il frutto delle politiche e delle non politiche di trasporto di questi anni, viaggia su gomma, quindi sui TIR. Le difficoltà dell'autotrasporto - voglio dirlo agli illustri senatori dell'opposizione, che ho attentamente ascoltato,

dall'altro alla grande frammentazione del settore e alla carenza di infrastrutture, che genera una congestione del traffico doppia rispetto alla media europea; inoltre, vi è la grande difficoltà a fare sintesi tra la committenza e l'eccesso di domanda, che si trasforma in una rappresentanza associativa di ben 13 sigle, e l'enorme difficoltà nell'applicare le norme che Governi e Parlamenti hanno dato al settore negli ultimi quarant'anni. Come ha notato il bravissimo senatore Mura, hanno lavorato nella gestione di questo comparto importanti esponenti della politica italiana: da Signorile a Bernini, a Burlando, a Bersani, a Treu, a Uggé. Il risultato è quello che noi ci siamo trovati all'inizio della legislatura. Tra i firmatari della mozione n. 451 vi è un senatore, il caro amico Sangalli, del quale ho apprezzato l'intervento, che ha partecipato parecchie volte, nella sua esperienza associativa, ai tavoli del settore, e potrà confermare la difficoltà a trovare sintesi in questo comparto. Vede, senatore Sircana, non è un problema di schiena dritta.

che durò quasi tre giorni e che costò la perdita di 4 miliardi di produzione al nostro Paese; non risolse alcun problema dell'autotrasporto e diede vita a una serie di impegni del Governo di allora che non trovarono l'approvazione da parte del Parlamento. dice lei, la schiena dritta, far proclamare lo sciopero, non ha risolto di una virgola i problemi del Paese; anzi, ce li ha consegnati in modo aggravato nella fase successiva.

noi possiamo lavorare e condividere una serie di punti, ragion per cui, da questo punto di vista, è quanto mai opportuno il rinvio

a questo Governo è toccato gestire l'autotrasporto più difficile d'Europa, nel Paese che ha meno infrastrutture d'Europa d'Europa e che, territorialmente, è il più arduo da gestire d'Europa; in quel Paese che, come diceva Cavour, ha la difficoltà, per raggiungere i mercati dell'Europa - il più grande mercato di consumo del mondo - di attraversare le Alpi. A questo Governo è toccato gestire questo settore dell'autotrasporto in queste condizioni difficili, in una legislatura che, dal punto di vista economico, è la più difficile del dopoguerra.

poteva disporre di risorse che oggi non ci sono. Noi invece, nella crisi economica peggiore degli ultimi cento anni,

senza un giorno di sciopero, senza far pagare e ricadere le difficoltà di questo settore, come è capitato in tutti gli altri Paesi d'Europa con il blocco dei TIR, sull'economia del Paese, danneggiandolo ulteriormente e producendo un danno economico e sociale. questa sia schiena dritta, ma credo che sia stata capacità di gestione. Così come abbiamo gestito l'economia con l'allargamento della cassa integrazione in deroga: abbiamo gestito una fase sociale difficilissima in questo settore. Capisco che il

io, che invece vi ascolto per cercare di capire cosa posso fare di meglio oggi, domani e dopodomani nell'attività di governo a favore del settore dell'autotrasporto e dell'economia italiana, ascolto le vostre proposte, ma

Non è aumentato il costo del trasporto, e noi abbiamo gestito l'economia senza farle pesare il costo di un blocco del Paese, come sarebbe accaduto se non avessimo chiuso quella vertenza. Ma in questi anni abbiamo fatto qualcosa di più, ed io vorrei che il Parlamento italiano e i miei amici senatori dell'opposizione lo valutassero un po' meglio. In questi anni difficili di scarsità di risorse abbiamo lavorato sull'intermodalità come da nessuna altra parte d'Europa. Noi abbiamo salvato e sbloccato le risorse dell'*ecobonus* per le autostrade del mare, frutto di una legge del 2002 del precedente governo Berlusconi che l'Europa approvò soltanto cinque anni dopo. Quelle risorse sono state tutte impiegate a favore delle autostrade del mare. Abbiamo fatto di più, merito di questo governo e della maggioranza che ci ha appoggiati: quella legge importante e innovativa, che prevedeva per tre anni l'incentivo a chi spostava il TIR dalla strada al mare,

proprio per insistere su questa modalità, stante la situazione difficile delle infrastrutture italiane, abbiamo prorogato in questa legislatura gli incentivi per le autostrada del mare. Tant'è vero che l'Europa ha definito la nostra - uso il termine italiano - la migliore pratica di intermodalità d'Europa. Dovremmo esserne tutti fieri, perché in fin dei conti, al di là di un voto, che può essere espresso per una serie di motivi, tutti abbiamo condiviso e condividiamo questo

appiccicati a quell'errore storico, che fa sì che oggi la nostra situazione di infrastrutture stradali è del 40 per cento inferiore al resto dell'Europa; il costo della congestione del traffico è pari al doppio rispetto alla media europea,

non sono stati inventati in questa legislatura. Quando siamo arrivati in questa legislatura, lo Stato spendeva per l'autotrasporto 500 milioni di euro: 300 milioni nel bilancio strutturale dello Stato e 200 milioni come manovra finanziaria.

abbiamo guadagnato a gestire in questo modo la politica dell'autotrasporto. Ad oggi, a tre anni e mezzo dall'inizio della legislatura, il costo del trasporto italiano non è aumentato di una virgola.

riprendendo l'intervento del senatore Cicolani, la liberalizzazione votata nel 2005 purtroppo, nei due anni del Governo precedente, non fu regolata, in quest'Aula il Governo, nella persona del ministro Bianchi, all'inizio del 2007, chiese la proroga per i termini della regolazione di quella liberalizzazione che non venne compiuta nei due anni di quel Governo. Non solo, in quei due anni non si completò il piano della mobilità. Ma quelli erano anni in cui l'economia cresceva, in cui c'erano risorse da utilizzare.

Marco Filippi, che è veramente un pezzo di politica industriale, è scritta a pagina 83 del Piano nazionale della logistica.

ridurre il costo del lavoro per gli autisti dipendenti delle società strutturate, che sono quanto di meglio abbiamo nella nostra politica dei trasporti e che dobbiamo difendere. Non potendo fare altri interventi che riducano il costo del lavoro, abbiamo scelto quella strada.

che lavorano in tutta Europa, competitori a livello internazionale sul sistema trasportistico, che sono il nostro fiore all'occhiello - rischiano di delocalizzare per andare a cercare un minor costo del lavoro allo scopo di competere con i nuovi Paesi entrati in Europa, tutto e subito. e subito. Sicuramente potevamo fare di meglio. Ma vorrei soltanto far rilevare che abbiamo gestito, nei tre anni peggiori, dal punto di vista economico, degli ultimi cento anni,

vi garantisco che quello dell'autotrasporto (come può certificare il senatore Sangalli), con 13 sigle che vi partecipano e che hanno in mano un'arma di lotta che nessun altro ha, è il più complicato e difficile.

dall'altro garantiscono la sicurezza stradale e, poiché dovranno essere individuati negli accordi di settore, portano alla riapertura del dialogo, che negli ultimi anni è mancato, tra la committenza e l'autotrasporto nei vari settori, perché ogni settore ha le sue specificità e diversità. conclusione, consegno agli atti una serie di documentazioni per rispondere sia al testo della mozione che all'intervento in Aula del senatore Marco Filippi per quanto riguarda la questione dei pedaggi autostradali.

negli incidenti dei mezzi pesanti in Italia nel quadriennio 2005-2008 è stato di 5,3 persone ogni milione di abitanti, un valore tra i più bassi in Europa. Europa. La graduatoria vede l'Italia all'ultimo posto, la Slovenia al penultimo, il Regno Unito al terz'ultimo, la Germania al quart'ultimo, i Paesi Bassi al quint'ultimo, insieme alla Svezia, e poi alla Francia. Questa è una tabella EUROSTAT che consegno agli atti, così come

Il valore di questo documento di questo documento è reso straordinariamente importante dal fatto che è stato firmato da tutte le associazioni dell'autotrasporto. Questo documento certo non ha valore di norma, però è un pezzo della politica industriale del settore dell'autotrasporto che tutte le associazioni dell'autotrasporto, che hanno firmato l'accordo che ha poi prodotto la legge n. 127 del 2010, hanno firmato e sottoscritto.

costa 295,66 euro l'anno, mentre in Europa la media è di 114 euro. Oltre a questo, chiudono i rubinetti del credito: c'è una stretta

questa situazione in Italia è ampliata perché non esiste vigilanza. Io presenterò una proposta di legge per sciogliere la Banca d'Italia che, invece di controllare l'operato dei banchieri, ci va a braccetto. Noi abbiamo la signora Tarantola che era amica, per esempio, di uno dei furbetti del quartierino. Il Governo non può fare orecchie da mercante.

queste situazioni perché, ripeto, questo è un grande Paese. Qualcuno vorrebbe celebrare i funerali dell'euro: qualcuno si deve opporre. I banchieri non possono andare a celebrare i funerali dell'euro negando, con la stretta creditizia, il credito a chi ne ha bisogno e a chi lo